Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228 «Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,

Presidente, avendo verificato i contenuti del maxiemendamento, non possiamo non ribadire quanto da noi già affermato durante la discussione. Troviamo l'ultimo provvedimento presentato dal Governo carente sotto il profilo politico, e contraddittorio sulla distribuzione territoriale e sociale dei sacrifici. Non ci convince il ricorso sistematico all'iniquo meccanismo dei tagli lineari. Valutiamo un peso della manovra eccessivamente sproporzionato su enti locali e Regioni, con l'aggravante che all'interno delle stesse si ritrova una sperequazione fortissima tra Mezzogiorno e resto del Paese. Cito i dati: il peso per le Regioni a statuto ordinario del Sud sarà di 211 euro *pro capite*, contro i 194 del Centro e i 129 del Nord. Del resto, abbiamo la sensazione che l'entità di questa manovra non sia sufficiente ad affrontare i problemi che la crisi pone al Paese. Nutriamo il sospetto che si dovrà reintervenire per ritoccare ancora i conti di un'economia nazionale che presenta fondamentali sempre più precari. Ed invece, oggi, siamo chiamati a votare fabbisogni sottostimati e insufficienti. Forse lo si fa perché manca il coraggio di presentarsi al Paese dicendo che non era vero che la crisi era solo psicologica, frutto di disinformazione, e che bisognava restare ottimisti perché mezza Italia viaggiava in corsia di sorpasso. Di certo, finiamo per affrontare una manovra che avrebbe avuto un evidente bisogno di reperire maggiori risorse, come quelle necessarie per sostenere crescita e domanda interna ed evitare, così, di licenziare un provvedimento sostanzialmente depressivo. In tal senso basta vedere come sono state trattate quelle circa tre milioni e mezzo di famiglie legate al pubblico impiego (magistrati, professori, forze dell'ordine, medici, infermieri, vigili del fuoco, ricercatori ), che rappresentano, insieme agli imprenditori, il motore di una moderna società. Ma, allora, perché non inserire almeno le risorse necessarie allo sviluppo e alla crescita? Perché non evidenziare che la realtà economica e finanziaria del nostro Paese richiede sacrifici concreti e significativi al punto che forse qualcuno dovrà iniziare a ripensare uno stile di vita troppo fondato su debiti e consumi? Probabilmente perché in quel caso si sarebbe dovuta raccontare la verità rispetto al modello che ci propina questo Governo. Nello scenario mondiale noi abbiamo assoluta necessità di rafforzare alcuni nostri punti di forza. Ad esempio, quelli che ci derivano dalla comune appartenenza al nostro Paese, nella sua unità, oltre che nella sua unicità, oppure, come sollecita spesso il Presidente della Repubblica, quelli che ci consegna la comune appartenenza all'Europa unita. Solo in questo modo si possono affrontare anche gli effetti negativi della globalizzazione - *humus* dentro cui pure si alimenta ed esplode la crisi -, affrontandola anche per i suoi risvolti positivi, per esempio attraverso la semplice constatazione della fuoriuscita dalle condizioni di povertà di qualche miliardo di essere umani, e non solo demonizzandola, magari al fine di alimentare quei sentimenti di paura e di egoismo sui quali costruiscono il proprio consenso determinati movimenti politici locali e divisionisti. Di sicuro non ci possiamo presentare divisi. Altro che diritto alla secessione! Altro che quote latte o Ministeri sminuzzati di qua e di là! Questa insufficiente e modesta manovra, contestata in tutta Italia, dimostra quanto meno alcune cose inconfutabili: non ci sono le risorse per pensare oggi al federalismo e, soprattutto, questo tipo di federalismo non serve al Paese. Il Ministro dell'economia questo lo sa bene, ma, consapevole che su questo imploderà definitivamente l'attuale maggioranza, deve tenerlo nascosto, in particolare agli elettori della Lega Nord, e minimizzare. Per questo non è servito a nulla provare a dare una mano. Noi lo abbiamo fatto attraverso 26 emendamenti alla manovra pensati per affrontare nodi strutturali e recuperare oltre 5 miliardi di euro. Ma non si è voluto mettere mano ai costi della politica, al finanziamento pubblico ai partiti, alla riduzione delle Province oggettivamente inutili. Non citerò tutti gli emendamenti: mi accingo Solo su un punto siamo riusciti a far ragionare la maggioranza: mi riferisco all'emendamento sulla microinvalidità e la possibilità di ridurre le tariffe ai cittadini da parte delle assicurazioni. Capirete tuttavia che non basta un solo emendamento per votare la fiducia. Rimaniamo dell'idea che questa manovra economica sia senza una "utile" visione politica, sia iniqua e priva di quegli interventi strutturali di cui avrebbe bisogno il Paese. Ed è per questo, oltre che per la semplice constatazione che noi non sosteniamo questo Governo, che annunciamo il voto contrario di Alleanza per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo*

cogliendo la necessità di questi interventi rigorosi, aveva immaginato alcuni emendamenti che traevano le risorse per il sostegno alle fasce sociali più deboli, per esempio prevedendo un limitato incremento della tassazione delle rendite finanziarie, portandolo oggi ad una media del 15 per cento, per poi salire gradualmente nel tempo verso la media europea. Questo avrebbe consentito di ricavare una quantità di risorse non non molto consistenti, ma sufficienti ad intervenire sulle aree più deboli, evitando interventi troppo drastici sul sul sistema di spesa pubblica che, è vero, ha delle aree di improduttività e di spreco, ma spesso sostiene non solo la domanda interna ma anche la tenuta sociale del nostro Paese. Il Governo ha fatto una scelta diversa, quella di tagliare molto sul pubblico impiego, sulla scuola, sulla sanità, sulle Regioni e gli enti locali con qualche difficoltà di relazioni istituzionali (ne abbiamo preso atto), ed anche con qualche ripercussione - immaginiamo - sulle famiglie e sui consumi, che possono non incoraggiare la ripresa, di cui si parla, ma che non viene colta quando non viene percepita in modo serio dagli osservatori e neanche dai cittadini. Non riteniamo che un tipo di taglio così drastico sul sistema di spesa pubblica attraverso il meccanismo dei tagli lineari sia il più il più opportuno, anche se è una scelta che il Governo ha sostenuto con grande convinzione e con grande rigore, misurando anche la sua capacità di tenuta nel rapporto con la maggioranza e con le forze sociali. Ebbene, io credo che in queste scelte, signor Ministro, il Sud paghi un prezzo molto alto. Nei vari interventi complessivi di recupero delle risorse, compreso quello sulle risorse stanziate per investimenti non ancora impegnate, l'operazione di di dragaggio che il Governo compie priva il Sud di molte possibilità. Ciò avrebbe dovuto determinare nel Movimento per le Autonomie la scelta di contrastare e di non votare questa manovra, se non avessimo intravisto, dopo tanto tempo, una prima risposta positiva a un problema reale di un territorio importante del nostro Paese, come la Sicilia. Abbiamo posto in modo trasparente il problema della sofferenza e della drammatica condizione del precariato, abbiamo sottolineato il rischio gravissimo di tensioni sociali, se non si fosse trovata una soluzione equa e trasparente

Poiché avevo detto in Commissione, a nome del Movimento per le Autonomie, che ove questo problema fosse stato risolto in modo soddisfacente, per quanto non definitivo, il Governo avrebbe avuto il nostro consenso, il nostro voto, richiamandomi alla vecchia regola, che vorrei anche il Governo osservasse

Signora Presidente, signori Ministri, l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo su un provvedimento che avrebbe dovuto coinvolgere il Parlamento e spiegare all'intero Paese l'utilità di misure per l'uscita da una delle più gravi crisi economiche non è ‑ come ha detto il presidente Berlusconi giorni fa ‑ un atto di arroganza o, come vuole farci credere, un atto di coraggio. È semplicemente un atto di viltà politica. Non è forse un atto di viltà politica che soltanto due mesi fa il Ministro dell'economia abbia smentito pubblicamente la necessità di una manovra finanziaria, parlando tutt'al più di un aggiustamento di poco conto, mentre sapevamo che già a novembre dello scorso anno il Consiglio dell'Unione europea con l'ECOFIN aveva sollecitato l'Italia a correggere e non oltre il 2 giugno, e a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo? Non è forse un atto di viltà politica che il Presidente del Consiglio, che avrebbe dovuto senza esitazione, come succede in qualsiasi sana democrazia occidentale, parlare alla Nazione e spiegare i sacrifici che ad essa si chiedevano, non abbia avuto il coraggio di metterci subito la faccia, dato che ancora un mese fa continuava a prenderne le distanze, dichiarando: «Questa finanziaria io non l'avrei mai fatta»? Non è forse un atto di viltà politica, che - fuggendo o rinviando ogni confronto con le altre istituzioni continui a nascondere dietro lo stucchevole ritornello che la manovra è richiesta dall'Europa, facendo quasi intendere che, se dipendesse dal Governo, di questa manovra si potrebbe anche fare a meno? Il Governo si è ben guardato dallo spiegare agli italiani che l'Unione europea chiede soltanto di mettere a posto i conti. Come farlo, come distribuire l'onere, a chi chiedere i sacrifici sono scelte che spettano alla classe dirigente di ogni Paese e che ogni classe dirigente responsabile e degna di questo nome sa come difendere e spiegare al proprio Paese. Non è forse un atto di viltà politica, nascondendosi dietro l'alibi di emendamenti parlamentari firmati alla cieca, di errori di penna, di sviste e di refusi, aver tentato sino all'ultimo di introdurre condoni fiscali ed edilizi, attacchi alle garanzie contrattuali, limiti ai diritti previdenziali acquisiti, mortificazioni all'assistenza sociale delle invalidità? Diamo onore alla Lega! Almeno loro hanno avuto il coraggio di sostenere fino alla fine la vergognosa sanatoria per i 67 allevatori che si rifiutano di pagare le multe rateizzate delle quote latte, nonostante gli accordi sottoscritti in Europa. Diamo onore alla Lega! Almeno loro sono riusciti ad ottenere, con il silenzio assordante di questa maggioranza, la proroga ulteriore di pagamenti per sanzioni, già dilazionati con una legge dello Stato a 12, 15, e 30 anni. Ma diamo onore, signor Ministro, anche ai terremotati d'Abruzzo, la mia terra, che per modificare l'articolo 39 di questo decreto e poter riaffermare il loro diritto, già applicato ad altri, di una proroga dei tributi per soli 10 anni, non per tutti e in parte, hanno saputo con dignità e senso civico affrontare i respingimenti delle forze dell'ordine schierate da questo Governo. Signor Ministro, in un Paese non lontano dal nostro, in Germania, è stato scritto un piccolissimo numero nella Costituzione: 0,35 per cento nel rapporto defìcit*-*PIL come soglia massima da raggiungere entro il 2016. Il che significa, da qui ad allora, risparmiare ogni anno 10 miliardi di euro, chiedendo al Paese, a tutto il Paese, una prova di verità, di realismo, di rigore e soprattutto di responsabilità, rivolta a tutti. È infatti infatti già stata determinata l'imposta sulle imprese interessate al mantenimento di 17 centrali nucleari e stanno definendo nel dettaglio una tassa sulle banche. Anche il nostro Governo vuole cambiare la Costituzione, ma lo vuole fare all'articolo 3, perché i cittadini non sono tutti eguali davanti alla legge, cosicché il Parlamento ha impiegato due terzi del suo tempo su emendamenti bloccaprocessi, sul processo breve, sulla legge del legittimo impedimento, sulle modalità di trasformazione del lodo Alfano in lodo costituzionale, sulle modalità di risolvere i contenziosi tributari e civilisti delle società del Capo del Governo. Anche il nostro Governo vuole cambiare la Costituzione, all'articolo 4, come ha ricordato il suo collega ministro Brunetta, perché, in un Paese di cassaintegrati e precari, promuovere le condizioni del diritto al lavoro non è più un cardine essenziale della nostra società. La vuole cambiare anche all'articolo 21, perché manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e lo scritto deve essere assoggettato ad autorizzazioni o censure. Questa manovra finanziaria è l'ennesima menzogna che si sta propinando al Paese. Se resta così, in assenza di riforme strutturali e giustizia redistributiva, non potrà stabilizzare i conti pubblici. Infatti, nel momento in cui lo stesso Governo ne riconosce il carattere restrittivo e recessivo, ammettendo un impatto negativo sulla crescita economica pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2010-2012, sa bene che per riportare il debito sotto controllo, fermo restando il tasso di interesse pagato sul debito pubblico, il livello di inflazione e gli oneri derivanti dall'invecchiamento della popolazione, con una ipotetica con una ipotetica crescita del saldo primario allo 0,8 per cento, manovre correttive sui nostri conti andrebbero varate per cinque anni di seguito. Sono di pochi giorni fa i dati del debito pubblico italiano, che ha raggiunto il nuovo record di 1.827 miliardi di euro: 15 miliardi in più rispetto ad aprile e 65 miliardi in più in cinque mesi. Ha ragione il ministro Tremonti quando afferma che «la rilevanza del debito a livello nominale è di importanza fondamentale, ma non esclusiva». allora può ancora aiutarci e potrà ripararci dal rischio di attacchi speculativi sui titoli del nostro debito da parte degli intermediari finanziari?

Da cittadini europei chiediamo quale credibilità, davanti al consesso internazionale, possiamo dare ad un Governo che da due mesi lascia vacante, in un momento di grave crisi economica, l'importante ruolo di titolare del Ministero per lo sviluppo economico perché bloccato da lotte di correnti e di fondazioni. Quale credibilità possiamo dare ad un Governo in cui soltanto ieri si è dimesso il Sottosegretario all'economia, perché su di lui pende una richiesta di custodia cautelare per partecipazione ad associazione a delinquere di stampo camorristico? Quale credibilità possiamo dare ad un Governo che nel quotidiano consente il prosperare di cosche e cricche e, nel loro frantumare la dimensione pubblica in una miriade di centri di interesse, riafferma la prassi consolidata in cui sfocia l'avversione per ciò che è legalità, per ciò che è il sentimento civico, per ciò che è il senso dello Stato? In questa manovra manca più di tutte una cifra essenziale: la cifra etica, quella dell'equità, della giustizia redistributiva, della solidarietà, che è il vero collante della tenuta e della coesione sociale del nostro Paese. *(Richiami del Presidente)*. Non c'è nessun articolo, comma o capoverso in cui si parli di giovani; eppure, mai prima d'ora la crisi aveva colpito così tanto i nostri giovani, mettendo a rischio un'intera generazione. O meglio, si parla di loro nel congelare le assunzioni, ridurre le quantità di contratti a termine, falcidiare la formazione professionale. Non c'è nessun articolo, comma o capoverso, che ci parli della famiglia, in un Paese in cui vivono 975.000 famiglie...

Non c'è nessun articolo, comma o capoverso in cui si parli di imprese, in un Paese in cui la mortalità imprenditoriale sta colpendo anche le Regioni più ricche del Nord-Est, tranne all'articolo 42 sulle reti

costringendo ancora una volta il Parlamento a subire una scelta senza poterla neanche discutere. Non è un atto di coraggio, come dice il Presidente del Consiglio, né un atto di forza. La fiducia è solo l'ennesimo atto di debolezza per tirare a campare, nascondendo i dissidi interni; è figlia della soggezione politica, anzi della schiavitù, a una piccola parte del Paese. Per essere chiari fino in fondo: quella che votate oggi non è la fiducia al Governo ma un atto di sottomissione al padrone del Governo, che porta il nome di Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Da subito ci siamo resi disponibili a collaborare nell'interesse del Paese, perché la crisi economica internazionale, unita alla sottovalutazione degli scenari negativi della nostra contabilità pubblica, impone una rapida quanto efficace inversione di rotta nella gestione del bilancio dello Stato. Da opposizione responsabile e non disfattista quale siamo, vi abbiamo chiesto di scrivere insieme in Parlamento un provvedimento efficace per risanare in profondità l'economia italiana, convinti come siamo che l'Italia ha bisogno di riforme a cominciare dal sostanziale miglioramento della qualità della spesa pubblica, presupposto indispensabile per la crescita. Purtroppo, avete dimostrato di non avere né il coraggio né l'umiltà necessari per affrontare l'emergenza economica. Siete prigionieri della vostra ostinata presunzione d'infallibilità e di autosufficienza. Questa vostra spocchia vi fa scadere nell'autolesionismo, rinviando decisioni che sono indispensabili per mettere in sicurezza il Paese dalla crisi, irrobustendolo con riforme strutturali di medio e di lungo periodo. La crisi poteva rappresentare un'occasione per rinsaldare l'interesse nazionale, migliorando al contempo la qualità della nostra vita politica ed istituzionale. State invece approvando un provvedimento che, seppur in linea con le indicazioni europee, rinvia a tempo indeterminato quei necessari aggiustamenti strutturali di entrata e di spesa che ci rendono più forti e competitivi. In altri termini, siete riusciti a trasformare una manovra economica oggettivamente inevitabile in un provvedimento di corto respiro, la cui idoneità ad incidere strutturalmente sui conti pubblici non è certa e che, peraltro, non offre alcuno stimolo concreto sul fronte della domanda. Eppure la condizione del Paese è nota: nel biennio 2008-2009 il PIL è sceso di 6,5 punti, cioè quasi metà della crescita che si era avuta nei dieci anni precedenti.

sulle ore lavorate nell'industria è salita al 12 per cento alla fine del 2009. L'occupazione è diminuita dell'1,4 per cento ed il numero di ore lavorate del 3,7 il 1994 ed il 2007 il rapporto tra debito pubblico e PIL era diminuito di 18 punti percentuali. Nel biennio di recessione 2008-2009 il rapporto è cresciuto di ben 12 punti percentuali, collocandosi al 115,8 per cento. L'esplosione della crisi greca, poi, ha operato come la benzina sul fuoco. A fronte di questa situazione di disagio crescente, la domanda che ci poniamo e che vi poniamo è se questa manovra è risolutiva dei problemi o se, viceversa, si colloca nel solco della continuità con i precedenti provvedimenti del Governo i quali, piuttosto che affrontare la crisi, si sono limitati ad esorcizzarla. Bisogna riconoscere che questa manovra ha dimensioni rilevanti perché opera una correzione dei conti di circa 25 miliardi di euro in tre anni, con molteplici interventi, sia sul versante della spesa, che sul versante delle entrate. Non abbiamo difficoltà a giudicare positivamente le disposizioni che combattono l'evasione fiscale. La prima vera novità della manovra, infatti, è proprio questa. Il Governo ha cambiato rotta, abbandonando definitivamente il populismo dell'insofferenza fiscale che vede lo Stato come un inutile succhiatore di sangue dei contribuenti. Tuttavia, non è certo che le norme antievasione contenute nella manovra siano idonee a garantire, nel breve periodo, l'effettivo conseguimento dei risultati previsti e contabilizzati sul versante delle maggiori entrate per lo Stato. Sul versante della spesa, la manovra incide massicciamente sul pubblico impiego. Gran parte delle misure adottate ha però un'efficacia di breve periodo, sicché il pericolo che corriamo è che, scaduti i tre anni di validità del blocco degli aumenti contrattuali, si assista ad una rinnovata crescita della spesa che pregiudichi i risultati conseguiti nel breve periodo. Lasciamo stare i danni in alcuni settori strategici, come la scuola, per non parlare delle forze dell'ordine e dell'intero comparto sicurezza completamente saccheggiato dalla manovra. Al comparto sicurezza sono sottratte anche quelle somme che in passato gli erano state riconosciute per la sua specificità e per il rinnovo del contratto di lavoro, con l'aggiunta della beffa delle promozioni senza aumento della retribuzione, che inaugurano anche in questo specifico settore della pubblica amministrazione la giungla retributiva, con personale che a parità di grado percepisce stipendi diversi. Però i soldi per rifinanziare le coreografiche pattuglie miste di militari e forze di polizia li avete trovati, e vi siete inventati un non meglio precisato fondo perequativo per il personale del comparto, che non ha alcun senso se non quello di elargire qualche mancia senza criterio. Come tutto ciò potrà incidere negativamente sul morale e sulla produttività degli operatori della sicurezza è facile prevederlo. La politica dei tagli lineari nei Ministeri, poi, senza alcuna verifica delle concrete sacche di inefficienza e di spreco settore per settore, rischia di produrre, allo scadere dei tre anni di vigenza della manovra, effetti di rimbalzo della spesa fortemente pregiudizievoli delle correzioni previste. Giudichiamo positive quelle disposizioni che innalzano l'età pensionabile, perché vanno tutte nella giusta direzione del riequilibrio strutturale dei conti pubblici previdenziali, compresi i refusi. A tale riequilibrio non corrisponde però una politica di sostegno ai giovani. La crisi economica ha aggravato le loro condizioni di precarietà nel mercato del lavoro. Secondo la Banca d'Italia, nella fascia di età tra i 20 e i 34 anni la disoccupazione ha raggiunto mediamente il 13 A fronte di questa condizione permanente di svantaggio, non vi è alcuna politica governativa che inverta la rotta anche attraverso il ricorso ad incentivi fiscali e contributivi all'occupazione giovanile. Eppure noi di proposte in tal senso ve ne abbiamo fatte tante durante la discussione parlamentare della manovra. Non ne avete voluta prendere alcuna in seria considerazione e avete sprecato quel poco di disponibilità economica residua in mance e mancette clientelari. Come definire, ad esempio, i soldi sprecati per la mini-naja, che invece potevano finanziare parte degli incentivi alle imprese che assumono giovani fino ai 30 anni? Questo Governo non ha una politica per i giovani e neanche un Ministro che sia messo nelle condizioni di occuparsene seriamente. La manovra continua ad ignorare la famiglia, soprattutto quella monoreddito e con più figli a carico, che esce ancora più povera dalla correzione dei conti pubblici. La manovra inoltre non colpisce quanti speculano sui risparmi delle famiglie italiane. La vicenda delle quote latte poi è una vergogna che offende gli agricoltori onesti del Nord e del Sud del Paese, che stanno sul mercato in condizioni difficilissime. Questa manovra è piena di marchette padane intollerabili e vergognose, a partire dalla mancata soppressione delle Province e dalla mancata fusione dei piccoli Comuni. Questa manovra chiude definitivamente e in senso assolutamente negativo la questione meridionale. Il Mezzogiorno non esiste più per il Governo. Lo dimostra l'inutilità delle zone a burocrazia zero e della finta fiscalità di vantaggio. Come possono le Regioni del Sud ridurre l'IRAP se il Governo con questa manovra taglia loro drasticamente i trasferimenti? Quali nuovi investimenti possono essere incentivati quando giustamente le Regioni meridionali devono velocemente rientrare dalla sovraesposizione finanziaria per i debiti accumulati soprattutto nel settore della sanità? La manovra maschera l'ennesima operazione in danno del Mezzogiorno, che riguarda la sottrazione dei fondi comunitari. Non basta la reprimenda del ministro Tremonti a coprire quest'operazione, perché, anche se è vero che la capacità di spesa delle Regioni è pessima, lo è pure, d'altro canto, quella dello Stato.

sopratutto quando lo fa dolosamente al solo scopo di sottrarre quelle risorse ai territori più disagiati per destinarle ad altri scopi, come è avvenuto in questi due anni, in maniera sistematica ed arbitraria. Questa manovra fa pagare il conto più salato a Regioni ed enti locali con i tagli operati direttamente sulle funzioni amministrative che esercitano per conto dello Stato. La conseguenza inevitabile è la contrazione dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese e l'aumento della pressione fiscale locale. È una manovra con cui lo Stato formalmente non mette le mani nelle tasche dei cittadini o le mette poco, ma le fa mettere a Regioni ed enti locali facendo aumentare la pressione fiscale. Il taglio alle Regioni non è l'anticipo del federalismo fiscale, ma la sua pietra tombale, perché tenta di porre un freno alla crescita incontrollata della spesa pubblica locale causata dal folle federalismo istituzionale introdotto con la riforma E mentre il Paese chiede di essere governato con efficienza, la maggioranza continua ad avvitarsi in dispute interne e faide di potere, senza capire che è arrivata l'ora di fare un'ampia operazione verità che porti a riforme strutturali e durature nell'interesse del Paese. Ci dispiace, ma non possiamo votare questo provvedimento perché è iniquo ed inadeguato rispetto ai gravi problemi del nostro debito pubblico. Il conto più salato lo pagano sempre le famiglie, le nostre forze dell'ordine ed i cittadini più bisognosi. Noi non possiamo accettarlo.

Non solo rischiamo di perdere i 44 miliardi di euro della *tranche* 2007-2013, se non saranno impegnati entro la fine dell'anno, ma addirittura, in ambito europeo, si parla di rivedere le politiche di coesione dopo il 2013. In buona sostanza, rischiamo di non prendere più neanche

La principale misura strutturale contenuta nella manovra è la riforma definitiva delle pensioni. È una riforma definitiva: semplicemente, in futuro non serviranno altre leggi, perché l'età pensionabile aumenterà automaticamente di quanto aumenta - come tutti ci auguriamo - la vita media. Di questo si è parlato poco o nulla. Sono state poste a pedaggio tratte di autostrada che ingiustificatamente erano pagate da tutti i contribuenti. Anche l'annosa questione dei lavoratori socialmente utili siciliani ha trovato una soluzione di buonsenso. Sappiamo benissimo che non è possibile lasciare a casa dall'oggi al domani 23.000-25.000 persone: anziché rifinanziare come tutti gli anni questa proroga, si è data la possibilità di farla, pagandola attraverso le economie di bilancio, con una soluzione di buonsenso. intervento strutturale e molto importante che è passato quasi sotto silenzio è il divieto di ripiano delle perdite delle aziende partecipate. Questa è davvero una misura strutturale importantissima: in questo modo chiuderanno centinaia e centinaia di carrozzoni, veri e propri stipendifici che, senza il ripiano automatico delle perdite da parte di Comuni e Province, dovranno portare i libri in tribunale. inoltre previsto l'accorpamento obbligatorio delle funzioni per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che, oltre a comportare un risparmio notevolissimo di costi per gli enti locali, garantirà servizi migliori ed efficienti.

Un altro importante taglio virtuoso è rappresentato dal divieto di sponsorizzazioni: finalmente non vedremo più Comuni o Province con bilanci in dissesto sponsorizzare addirittura squadre di serie A o di serie B.

Inoltre, c'è un'indagine in corso: finalmente si potrà arrivare alla verità su una questione complessa, che si trascina da anni, e si potrà mettere la parola fine anche su di essa. Un altro importante contributo della Lega riguarda la cosiddetta SCIA, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività. In sintesi, per aprire un'attività basterà notificarlo al Comune: finalmente si inizia a fare qualcosa di liberale anche in questo Stato. C'è poi lo sconto di oltre 200 milioni di euro sulla bolletta elettrica di famiglie e cittadini, che deriva dalla revisione del meccanismo dei certificati verdi. Oltre a questo, la Lega ha ovviamente proposto una serie di temi importanti dal punto di vista territoriale, che cito velocemente: la soluzione della questione degli alluvionati del Piemonte; il mantenimento del finanziamento di alcune strutture e infrastrutture praticamente già appaltate, quali la tranvia di Verona; la revisione di concessioni autostradali, come quella della A22 del Brennero, al fine di realizzare infrastrutture territoriali importanti; la soluzione della disputa sulle concessioni idroelettriche, che porterà benefici ai territori in cui insistono centrali idroelettriche. idroelettriche. Sappiamo però che la strada per giungere al pareggio di bilancio è ancora lunga, molto lunga, il buco fra entrate e uscite è ancora molto rilevante, strada è lunga, e poco il tempo a disposizione. Per fortuna, i decreti sul federalismo fiscale vanno avanti. A fine mese arriva quello, importantissimo, sui Comuni, che ha consentito di trovare un accordo importante con le amministrazioni La Lega ha ben chiaro che questa è l'unica via per coniugare tagli ed equità. Tutte le Nazioni avanzate sono organizzate in forma federale. La Lega vuole che non solo la Padania, ma l'Italia tutta, come ripete spesso il presidente Napolitano, rimanga agganciata al traino delle migliori Nazioni. *(Applausi Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, una parola di verità come esordio: non abbiamo mai messo in discussione né la necessità della manovra né la sua consistenza. Spero che affermarlo in questa sede così autorevole valga a fugare ulteriormente ogni dubbio e ogni strumentalizzazione. Abbiamo invece insistito, e continueremo a farlo, sul fatto che questa manovra è fortemente ed evidentemente iniqua e recessiva, destinata cioè ad impoverire il Paese di ogni prospettiva di crescita e di sviluppo. Poiché sono nell'età nella quale posso consentirmi di fare la persona saggia, vorrei guardare all'iniquità di questa manovra, alla sua straordinaria povertà di effetti nel tempo, al suo essere davvero così circoscritta all'oggi, a questo momento, parlando di una questione che non ricorre normalmente nei dibattiti parlamentari e che non ricorre, anzi, nelle parole della politica: è una questione riguardante i ragazzi e le ragazze di questo Paese. Non c'è una misura, in questa manovra, che riguardi le giovani generazioni, i ragazzi e le ragazze italiane. Eppure, nel 2009, il 63 per cento dei posti di lavoro persi è riconducibile a lavoratori dipendenti a termine, collaboratori a progetto: ragazzi e ragazze, normalmente. Nella fascia di età tra i 19 e i 29 anni, la perdita di occupati ha raggiunto le 300.000 unità, che corrispondono al 79 per cento della flessione complessiva e portano il tasso di disoccupazione giovanile in Italia al 25,4 che è più del triplo del tasso di disoccupazione nazionale e molto al di sopra di quello europeo (che è del 19,8 Secondo l'ultimo rapporto dell'ISTAT, dal 1983 ad oggi, si sono triplicati i ragazzi tra i 30 e 34 anni che vivono con i genitori, a testimonianza di una perdita di autonomia, ma anche di una perdita di fiducia senza precedenti nelle giovani generazioni italiane. Deteniamo il primato europeo per coloro che vengono definiti dall'acronimo NEET, cioè i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che sono al di fuori dal mercato del lavoro, fuori da ogni percorso di istruzione, fuori da ogni percorso di formazione.

ma mi fermo qui. Abbiamo presentato i nostri emendamenti a correzione parziale di questi drammatici dati e di questo *trend* ma, ovviamente, sono stati da noi presentati e discussi e da voi serenamente bocciati. bocciati. Né c'è traccia di una misura riguardante i giovani italiani nel maxiemendamento che sottoporrete, serenamente, al voto di fiducia.

non potrete così sfuggire, voi che siete, come me, padri e madri di figli privilegiati in questo Paese - privilegiati oltre ogni misura e per ogni ragione - al dato per ogni ragione - al dato essenziale che state venendo meno alla prima responsabilità di una classe dirigente, quella cioè di creare un'altra classe dirigente - dico di più: un popolo

E non c'è una misura sul Mezzogiorno. Avete vinto anche in Sicilia - lasciamo perdere quello che avete fatto dopo, in Sicilia - sull'onda del ponte sullo Stretto; ebbene - articolo 46 - gli unici soldi che ci sono, quei pochi che ci sono, sono destinati al MOSE: il resto, se guardiamo all'esperienza fatta in questi anni con i fondi FAS, li destinerete, serenamente, a spesa corrente. E questo, mentre alle donne italiane,

il mettere insieme il lavoro di cura della famiglia e dei figli ed il lavoro all'esterno, ed esse ringrazieranno vivamente, perché avete aumentato, fuori da ogni ragionevole previsione e fuori da ogni gradualità, di almeno cinque anni il termine per andare in pensione. Nessuna misura per la crescita, per gli investimenti, per lo sviluppo: i miei colleghi sono molto più bravi di me e ve lo hanno spiegato in ogni modo, in Commissione e in discussione generale. E allora vediamola, l'Italia che racconteremo dopo questa finanziaria. Cosa è accaduto in questi anni, quali sono le grandi riforme di cui il Governo Berlusconi può fregiarsi? La riforma sul federalismo: vero, ministro Calderoli? Quanto ci abbiamo lavorato, Ministro, per partire da un testo che noi non condividevamo e arrivare ad un testo che può rappresentare, e penso rappresenterà, in questa legislatura, l'unica occasione in cui le due parti, le opposizioni e la maggioranza, che si incontrano in quest'Aula, ma di più, le due parti del Paese, si sono parlate, si sono capite e sono arrivate ad un testo condiviso: con i tagli alle Regioni e ai Comuni, quel federalismo lì, che è coerente con i principi di sussidiarietà e solidarietà, che dà un'occasione al Mezzogiorno e alle sue classi dirigenti di mostrare responsabilità e buon governo, che dà prospettive di sviluppo e nuovi poteri ai cittadini e capacità di controllo sulle istituzioni pubbliche, è sepolto! Quello che torna - e per questo non fate una piega anche voi - è di nuovo la pistola in mano alle Regioni ricche: l'esecuzione stavolta è affidata alle Regioni ricche e ai cittadini delle Regioni più povere e in difficoltà toccherà una mattanza di diritti di cittadinanza. alla stessa riforma della pubblica amministrazione, un punto valeva a qualificarla come espressione di una politica moderna e avanzata, ed era quello di riorganizzare secondo efficienza, merito e produttività. Era l'unica parte che distingueva e dava un segno dell'innovazione alle politiche di questo Governo: l'avete ovviamente sospesa. *(Brusìo).* Capisco che i colleghi abbiano molti argomenti di cui interessarsi, ma preferirei avere un poco di silenzio, Presidente. Presidente Schifani,

Ma perché questa manovra? Il ministro Tremonti più volte, con la sua autorevolezza anche scientifica, e ancora ieri, ha detto tre parole, che condividiamo e sulle quali i nostri Governi precedenti hanno costruito politiche anche dure per il Paese: Europa, austerità, rigore. Bene, benissimo. Ma le parole non sono polisenso, ministro Tremonti: le parole hanno un solo netto significato. L'Europa non può valere per il saldo contabile e non valere per il Trattato di Lisbona; non può valere per il saldo contabile e non valere per il diritto allo studio, alla formazione e all'istruzione; non può valere per il saldo contabile e non valere per il lavoro e per i suoi diritti. Che Europa è? *(Applausi dal Gruppo PD).* E l'Europa, certo che dice bene: ha ragione. È ovvio che l'Europa dica bene, e che bene dicano tutti gli altri organismi che guardano a come l'Italia fronteggia una crisi economica e un debito pubblico spaventoso e una spesa pubblica fuori controllo - certo, fuori controllo - anche con voi: con con voi, anzi, il tasso di aumento della spesa pubblica è stato più vistoso e più consistente. Ma l'Europa non controlla le politiche. Cosa importa se per arrivare alla fine del mese affamate i figli piuttosto che rinunciare all'auto di lusso?

E allora, qual è il perché profondo di questa manovra? Ve lo dico in maniera brutale e anche molto sbrigativa. Il perché profondo è che in questa manovra non c'è alcuna strategia politica. Questa è una manovra contabile e, secondo me, non è fatta neanche tanto bene. Non siete stati neanche capaci di presentarla come si deve. Ministro Tremonti, le sue parole, austerità e rigore, risuonano con il carico di significato che hanno se sono insieme ad un'altra parola che pure lei ha usato, ed è quella che riguarda la giustizia: la giustizia della manovra, il fatto di gravare allo stesso modo e progressivamente, come dice la Costituzione, su chi ha poco o quasi niente e sugli sterminati patrimoni, sulle ricchezze e sulle rendite che da questa manovra non vengono tassati neanche per un euro.

a lei, ministro Tremonti, la prego di credermi. Allora avevano un significato. Ma dette oggi, mentre ci si squaderna sulle pagine di tutti i giornali, il sottobosco parassitario che cresce sotto il trono di chi intende regnare e non governare,

avrebbe difficoltà ad incontrare anche solo per un caffè, e che vengono accreditati per influire, condizionare, suggerire, telefonare, spingere, pressare sulle più alte cariche dello Stato, sui massimi dirigenti della magistratura italiana, sul Consiglio superiore della magistratura, sulla Corte costituzionale... PRESIDENTE. Senatrice ma non c'è cosa che non vada guardata politicamente in un contesto, e se devo guardare a questa manovra in questo contesto nel quale in due mesi due Ministri e un Sottosegretario di questo Governo sono stati davanti all'Italia costretti alle dimissioni per la vergogna, io le dico che, se non ci fosse da piangere, sarebbe davvero grottesco e ridicolo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentanti del Governo, questa manovra che giunge oggi al voto nell'Aula di Palazzo Madama è stata realizzata - lo vogliamo dire come prima considerazione - con un forte consenso delle parti sociali:

che hanno apprezzato questa manovra e questa è stata la dimostrazione di una forte coesione sociale. Vi è un partito del no (per carità, siamo in democrazia e sarebbe singolare se non vi fosse), ma i sì sono stati tanti, qualificati ed importanti. Vogliamo sottolinearlo proprio all'insegna della coesione sociale che il Governo e la maggioranza hanno cercato nel Paese. Con questa manovra, onorevoli colleghi, abbiamo evitato una crisi sociale interna

Noi abbiamo salvaguardato l'Italia anche con questa manovra e con gli interventi avviati negli ultimi due anni di governo da qualsiasi fattore rischio che ha colpito e sta colpendo - ripeto - altre realtà dell'Europa.

(fondi appositi per il comparto sicurezza-difesa, tutela piena delle invalidità, problematiche riguardanti vari territori della Repubblica al Nord, al Centro, al Sud e nelle isole, problemi concernenti il sistema produttivo) sono state accolte; a saldi invariati, sono stati apportati miglioramenti alla manovra in una sana, democratica e libera dialettica tra Parlamento e Governo. Anche di questo rivendichiamo con orgoglio il merito al nostro Gruppo, alla maggioranza e al Senato della Repubblica.

dovrebbe ricordarsi di spendere le cifre ingenti per la ricostruzione che, attraverso la Cassa depositi e prestiti ed altri strumenti, sono state appostate. Si chieda, ma si utilizzi ciò che doverosamente è stato messo a disposizione. Abbiamo incontrato Sindaci e Presidenti di Regione. Sappiamo che le Regioni dovranno fare la loro parte di sacrifici. Ieri sera mi è capitato di vedere in televisione un servizio su un ospedale della Regione Emilia-Romagna.

50 milioni di euro ed è già arrivato a costarne 500 milioni! Si facciano, dunque, meno sprechi sul territorio per dare più servizi ai cittadini: lo faccia lo Stato, lo facciano le Regioni e lo facciano le città! della sanità con questa manovra abbiamo garantito tutti i servizi essenziali ai cittadini. Non inseguiamo con nuove tasse la crescita della spesa pubblica: vogliamo contenere le dinamiche della spesa pubblica e non elevare il prelievo fiscale.

nuovi ed ulteriori strumenti per combattere l'evasione fiscale. Non vogliamo mettere più tasse per tutti, ma vogliamo far pagare le tasse a chi le ha ingiustamente evase: ci stiamo riuscendo anche con questa manovra e con la politica svolta negli ultimi anni dal Governo.

di semplificazione e di chiarezza: abolire leggi, abolire enti, abolire auto blu, ridurre i costi della politica, ridurre i rimborsi elettorali ai partiti, ridurre i costi di tutti gli apparati politici. Il presidente Schifani ha già annunciato che il Senato della Repubblica si uniformerà,

l'omogenizzazione stipendiale, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimenti, missioni e presenza qualificata in servizio. Tutto questo è negli emendamenti che abbiamo discusso ed approvato a tutela di prestazioni

quel fondo alimentato dai sequestri e dalle confische che ogni giorno vengono fatte alla camorra, alla mafia e alla 'ndrangheta. Continuiamo a togliere soldi al male per darli alla sicurezza e alla giustizia.

sono stati tagliati gli stipendi dei dipendenti pubblici del 2,5 per cento; in Italia, no. Si tagliano fino al 2014 15.000 posti di lavoro nel pubblico impiego; in Italia, no.

In Francia c'è una rivolta contro la riforma previdenziale; noi abbiamo realizzato una grande riforma delle pensioni, anche con questa manovra, senza un'ora di sciopero e con il consenso del Paese e delle parti sociali. Questo vuol dire lavorare per i giovani e per il futuro, presidente Finocchiaro. Non la retorica dei bamboccioni. La riforma delle pensioni.

si taglia la spesa pubblica del 25 per cento, si aumenta l'IVA, si alza l'età pensionabile. In Spagna hanno vinto la Coppa del mondo, ma aumentano l'IVA e il Governo Zapatero arriva ultimo nelle sue politiche economiche. In Spagna va meglio il calcio che la sinistra. Questa la verità dei numeri! I giudizi europei: i Ministri finanziari dell'Unione europea in questi giorni hanno detto che il Governo italiano ha agito conformemente alle raccomandazioni del Consiglio.

15 provvedimenti economici, salvato il credito, tutelato il risparmio privato, affermato in Europa nei giorni scorsi, grazie a Berlusconi e Tremonti, che il risparmio privato, in Italia che è forte, è un elemento da considerare nel bilancio degli Stati. Concludo ricordando due cose importanti, una della manovra e una contemporanea. La manovra, con la riforma delle pensioni, segna un momento di riforma strutturale del Paese. Abbiamo fatto riforme nella pubblica amministrazione, nella scuola e nella sicurezza; le faremo nell'università. Stiamo facendo le riforme strutturali del Paese. Mentre facciamo la riforma delle pensioni, a Pomigliano d'Arco la sinistra dei no ha perso e ha vinto quella responsabilità sociale che per la prima volta vede una produzione industriale, invece che andare dall'Italia all'estero, tornare dall'estero in Italia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Questo grazie a quegli operai che hanno votato sì e grazie al Governo, caro ministro Sacconi, che quell'intesa ha voluto e sostenuto.

garanzia per lo sviluppo e la crescita dell'economia. La nostra fiducia è convinta. Come sempre, agiamo in linea con l'Europa. Apriremo una stagione di crescita e di sviluppo.

Il Governo propone le seguenti quattro modifiche di mero coordinamento formale in relazione al maxiemendamento presentato: «Al disegno di legge di conversione, al comma 1-*bis*, dopo le parole "del comma 12 dell'articolo 12", inserire le seguenti: "del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78". n. 78". All'articolo 12, comma 9, il periodo che inizia con "All'onere derivante" deve intendersi come periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 12 e, nel medesimo periodo, sostituire le parole: "alla presente lettera" con le seguenti: "al presente comma". comma". All'articolo 12, comma 12-*ter*, i due capoversi che seguono devono intendersi come periodi aggiuntivi al predetto comma. comma. All'articolo 55, comma 2-*ter*, le parole: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94". *(PD)*. Signor Presidente, approfitto della presenza di questa proposta di coordinamento per segnalare un fatto, in verità piuttosto inquietante, che merita di essere conosciuto. Se voi, colleghi, leggete a pagina 43 del testo del maxiemendamento al nostro esame trovate una norma che in Commissione abbiamo scritto così con voto apposito, correggendo un errore che era stato compiuto precedentemente, nel coloro che esercitano l'attività di rivenditori di generi di monopolio devono conseguire una idoneità professionale - signor Ministro, si tratta dell'accesso ad un lavoro attraverso corsi che si faranno «sulla base di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'Organizzazione»

Dopo di che, nel testo finale della Commissione, compare un errore ulteriore: «le Organizzazioni maggiormente rappresentativa», al singolare. Sollevo nuovamente la questione e dico che bisogna correggere anche quell'aggettivo finale. Nel testo del Governo, signor Presidente, ricompare «l'Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa». Dubito che si tratti di un refuso ed invito il Governo ad inserire nella sua proposta di coordinamento anche la definitiva soluzione di questo problema, perché

Signor Presidente, volevo confermare che, nel corso dei lavori della Commissione, questo problema è stato preso in esame e concordemente,

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Hanno chiesto, e l'ho concesso, di votare per primi i senatori

con appello dell'emendamento 1.10000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78,

72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2,

per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009, aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni per l'anno 2009 presentate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2008. L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso aprile, con cui il MUD è stato modificato, non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. Si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato per la maggior parte dei soggetti obbligati, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, operativo dal mese di luglio 2010. Si tratta, come noto, di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Il SISTRI è stato disposto con la legge finanziaria del 2007 e successivamente istituito e disciplinato con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, relativi all'anno 2009, versamento che deve tenere conto delle riduzioni previste dalla legge finanziaria per il 2010. Tale termine, la cui scadenza annuale è fissata al 16 febbraio, era stato già prorogato al 16 aprile 2010 e ulteriormente prorogato con il presente decreto-legge per permettere l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione. Appare utile evidenziare che il termine prorogato è scaduto e che le disposizioni attuative citate non risultano essere state emanate al momento della redazione della presente nota. Viene quindi previsto che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e ad esse non si applicano le sanzioni civili previste dalla normativa, fermo restando l'obbligo in ordine al versamento di tali contributi per il 16 giugno. L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La dotazione della citata riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO2, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente. Si ricorda che l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2006, con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale il sistema di *emission trading*, dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni, pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO2 non restituita, fermo restando l'obbligo di adempiere, comunque, alla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. In mancanza di un'assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare tutte le quote di CO2 emesse sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario, soprattutto delle piccole e medie imprese, e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia. L'intervento recato dall'articolo 2 appare da mettere in relazione alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 aprile 2010, in cui sono state espresse preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote gratuite di emissioni di CO2. L'Autorità, nella medesima segnalazione ha ricordato inoltre, la mancata attuazione delle disposizioni recate all'articolo 2, comma 554, lettera *e),* della legge finanziaria 2008, che aveva previsto l'istituzione di un apposito Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da destinarsi all'acquisto di quote di CO2 con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti. Come noto, l'Unione europea, con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE, ha inteso anticipare la piena entrata in vigore dell'*emission trading*, previsto a livello internazionale solo dal 2008. Tale direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ha infatti previsto l'istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005, da affiancare all'*emission trading* previsto su scala globale dal Protocollo. La procedura prevista dall'articolo 2 può essere riassunta come segue: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dì C02 spettanti ai nuovi entranti rimasti esclusi dalle quote di riserva (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dei crediti per i citati soggetti esclusi determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall'articolo 10 della direttiva prima citata (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi. Come è noto, l'articolo 10 della direttiva citata prevede che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri mettano all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di stabilire l'uso dei dei proventi, utilizzando almeno il 50 per cento di questi per una serie di scopi ambientali, ivi indicati, di riduzione delle emissioni e di incremento dell'efficienza energetica. Relativamente alla liquidazione dei crediti, lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009. Il comma 18 dell'articolo 27 della citata legge prevedeva che, a partire dal 2011 (termine poi prorogato al 2012 dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135), il calcolo della quota obbligatoria di energia prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei certificati verdi, fosse effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'*import*, come attualmente previsto. Pertanto, veniva previsto che, a decorrere dal 2012, l'obbligo di immissione sarebbe passato dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o i venditori di energia.

I commi 4 e 5 demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2.

si trova oggi ad esaminare un decreto-legge di imminente scadenza (il 20 luglio) composto da due soli articoli ma che in realtà riguarda tre diverse materie: le emissioni di anidride carbonica, l'autotrasporto e il ciclo dei rifiuti. Stando ai comunicati del Consiglio dei ministri che possiamo trovare sul sito della Presidenza del Consiglio, il decreto in esame risulterebbe approvato il 30 aprile scorso, ma pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 21 maggio, sembra a causa di perplessità sollevate dalla Ragioneria dello Stato riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 2. Va inoltre rilevato come il decreto in esame risulti essere presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dello sviluppo economico *ad interim* (come è noto, entrambe le cariche sono ricoperte dall'onorevole Berlusconi, che ha sostituito il ministro Scajola, dimissionario, dal 5 maggio scorso). Un *interim* che era stato annunciato come brevissimo si prolunga dunque da oltre due mesi, per motivi evidentemente attinenti a problemi di assetto politico interno della maggioranza, ma ma che certo non giustificano il fatto di vedere un Ministero chiave come quello dello sviluppo ancora privo di titolare definitivo durante una grave crisi economica. Ciò premesso, si può entrare nel merito del provvedimento, precisando che gli effetti dell'articolo 1 si sono già esauriti nel momento in cui l'Aula del Senato ne inizia l'esame. l'articolo 1, comma 1, riguarda i tempi e le modalità di presentazione del modello di dichiarazione ambientale (MUD) da parte degli operatori del settore dei rifiuti. La proroga che esso dispone consente alle circa 600.000 imprese interessate di poter utilizzare ancora il MUD 2008 nell'imminente entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Ogni anno nel nostro Paese si producono quasi 150 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, dei quali il 10 per cento è classificabile come pericoloso. Con decreto ministeriale del 9 luglio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 di ieri, i termini per l'avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo dei rifiuti sono stati posticipati al prossimo 1° ottobre, con partenza unificata per piccole e grandi imprese. Il SISTRI, di cui bisognerà comunque verificare in corso d'opera le eventuali criticità, che peraltro stanno già emergendo, dovrebbe consentire il tracciamento elettronico totale del ciclo dei rifiuti, ed è bene che tale sistema entri velocemente in vigore senza più proroghe, risolvendo i problemi di onerosità che le imprese hanno segnalato. Del tutto eterogeneo è invece il contenuto dell'articolo 1, comma 2, che proroga il termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Tale norma nulla ha a che fare con la materia ambientale e contiene una clausola di non sanzionabilità nei confronti delle imprese che non abbiano provveduto al pagamento dei premi assicurativi all'INAIL secondo le scadenze previgenti, oppure che abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. In sostanza, tali imprese sono considerate per legge in regola sotto il profilo contributivo e non gli si applicano pertanto le sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000. A tali imprese dovevano essere destinate risorse derivanti dallo scudo fiscale ma, allo stato attuale, non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui verrebbero trasferite le risorse derivanti dallo scudo fiscale. Anche questa proroga, come quella sul MUD, è già scaduta mentre la esaminiamo e quindi è inemendabile; ma restano forti perplessità sia sul modo di legiferare con continui differimenti, sia sullo scudo fiscale e sui suoi miracolosi effetti, che ancora non si sono visti, se non per coloro che se ne sono avvalsi. Venendo all'articolo 2, che è l'unico che ancora dispiega i suoi effetti, dobbiamo rilevare come la scelta del Governo sia quella di assegnare a titolo gratuito quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti industriali a maggiore emissioni di gas serra entrati in esercizio dopo l'aprile 2009. È certamente vero che a quella data si era esaurita la «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione dì assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, con la conseguenza che si trovano scoperti tutti quegli impianti entrati in funzione successivamente. Tuttavia, non si vede e non si capisce perché l'onere dei 780 milioni di euro derivante da tale assegnazione non possa essere diversamente coperto. Infatti, dal 2013 partirà un sistema di aste per tutte le quote, comprese quelle finora assegnate Ricordiamo anzitutto che gli impianti interessati sono quelli per la produzione di energia elettrica, raffinazione, siderurgia, cemento, calce, vetro, laterizi, carta ed impianti di combustione con potenza superiore ai 20 megawatt. Si tratta quindi di grandi impianti, come quelli di Modugno e Civitavecchia, spesso appartenenti ad aziende altrettanto grandi che pure avrebbero potuto acquisire le quote sul mercato. Tuttavia dobbiamo prendere atto che l'Antitrust ha segnalato al Parlamento l'effetto distorsivo della concorrenza derivante dall'esaurimento anticipato delle quote gratuite, che determinerebbe un discrimine tra nuovi entranti e operatori già esistenti, i quali hanno già beneficiato dell'assegnazione. Il Governo Prodi aveva chiesto all'Unione europea di assegnare 230 milioni di tonnellate di quote, mentre ne furono concesse all'Italia circa 30 milioni in meno, più o meno quelle che ora vengono riassegnate gratuitamente. Per questo, nella precedente legislatura era stato previsto un Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare proprio alla riserva nuovi entranti, ma il Governo in carica lo ha praticamente azzerato, con il risultato che ora le imprese interessate vantano un credito complessivo compreso tra i 630 e i 756 milioni di euro: 477 milioni di euro per gli impianti entrati in funzione successivamente all'aprile 2009, cui si somma un importo stimato in 280 milioni di euro per gli impianti destinati ad entrare in funzione entro il 2012. Al suddetto importo complessivo vanno aggiunti gli interessi legali, per un totale stimato di circa 780 milioni di euro di finanziamento agli emettitori (anche grandi emettitori) di anidride carbonica. Poiché, stando al decreto-legge in esame, i proventi delle future aste vengono utilizzati per coprire tale spesa, quando la normativa comunitaria ci dice che essi dovrebbero essere destinati almeno per il 50 per cento per politiche a favore del clima, ridurre le emissioni, accrescere l'efficienza energetica, sviluppare le fonti rinnovabili, viene da domandarsi se l'onere derivante dall'articolo 2 non finirà col rendere più complicato il raggiungimento degli obiettivi comunitari «20-20-20», come indicati dalla direttiva n. 87 del 2003 e dalla direttiva n. 29 del 2009. Apprezziamo il fatto che alla Camera il Governo abbia assunto l'impegno a rispettare quegli obiettivi e vorremmo che altrettanto si facesse in Senato. A tal proposito, abbiamo presentato un ordine del giorno. Non è neppure chiaro il motivo per cui si preveda oggi l'abrogazione dei commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009, vale a dire il collegato energia dello scorso anno. Si tratta di una legge evidentemente molto sfortunata se ben due decreti-legge contemporaneamente all'esame del Senato la modificano in maniera rilevante a neppure 12 mesi dalla sua entrata in vigore: abbiamo infatti in corso di esame anche il decreto-legge n. 105, che cancella inspiegabilmente le incompatibilità per l'Agenzia nucleare. L'operazione relativa ai suddetti commi, nel suo complesso, si connette all'intervento sui certificati verdi contenuto nel decreto-legge sulla manovra appena approvata. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che, anziché intervenire con tagli ai finanziamenti per i piccoli-medi impianti concedendo contemporaneamente un beneficio rilevante per grandi impianti emettitori di anidride carbonica, sia ormai necessario ed urgente un intervento di riordino del sistema degli incentivi, per togliere di mezzo una volta per tutte le distorsioni del CIP6 per le fonti assimilate e dei certificati verdi, armonizzando la normativa italiana a quella comunitaria. Ci auguriamo che il recepimento della direttiva quadro europea entro la fine dell'anno sciolga questi nodi, che da tempo rallentano lo sviluppo delle fonti rinnovabili cosiddette pulite.

relativi alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con riferimento al 2009 e l'ulteriore proroga al 16 giugno 2010 del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL

è stato spiegato dalla maggioranza, si è resa necessaria in quanto non è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio di attuazione di una disposizione della legge finanziaria del 2010, che riduce i premi assicurativi per le aziende di autotrasporto di merci in conto terzi. Per tale ragione, lo stesso comma 2 dell'articolo 1 dispone la non applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge dì conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Vale la pena ricordare che alla proroga del MUD, in realtà, si è arrivati in modo sofferto dopo una serie di annunci e smentite, errori e ritardi. Finalmente il quadro normativo sembra ora completo e le 500.000 imprese tenute alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale possono tirare un sospiro di sollievo. Attesa l'esigenza di utilizzare anche per quest'anno il vecchio modello MUD per opportunità e per non gravare sulle imprese, si era stabilito, a parole, di prorogare il vecchio modello, ma di fatto non si provvedeva all'emanazione delle norme necessarie per realizzare tale esigenza. arrivati a ridosso della scadenza del 30 aprile 2010 nella più completa incertezza e confusione, sia da parte degli imprenditori, che delle Camere di commercio. Tornando al testo del decreto-legge in questione, l'articolo 2 reca misure urgenti in materia di assegnazione delle quote di anidride carbonica ai nuovi impianti entrati in esercizio. Il comma 1 richiama la definizione di «nuovo entrante», prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2006, che qualifica come «nuovi entranti» nel periodo 2008-2012 gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione. Risulta evidente, dunque, per quanto riguarda l'articolo 1, che si tratta di termini scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 giugno 2010; entrambi i differimenti si rendono necessari per la tardiva o la mancata emanazione di decreti del Presidente del Consiglio e perché, al mancato rispetto dei termini suddetti, sono connesse conseguenze di ordine sanzionatorio. Con riferimento all'articolo 2, in mancanza di un'assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese e sul mercato dell'energia elettrica, per gli inevitabili riflessi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia.

non vorremmo che la norma dell'articolo 2, nel prevedere l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, premiasse le imprese che superano i limiti di emissione, attribuendo loro una sorta di licenza ad inquinare, in contrasto con gli indirizzi normativi

altro non vuol essere che un sollecito al Governo perché dia immediata attuazione al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo adottato dal Governo nelle scorse settimane dopo il parere della Commissione ambiente, che in quella previsione è stato interamente recepito. Si tratta quindi di un semplice sollecito al Governo

presto diventare oggetto di un decreto istitutivo di area marina protetta. Questo è il contenuto dell'ordine del giorno, che spero il Governo voglia accogliere.

ad esprimere il parere sull'ordine del giorno

Esaminati, altresì, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando a valutare, quanto all'emendamento 2.3, la compatibilità della disposizione ivi prevista con le competenze regionali in materia di realizzazione degli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento all'eventuale incidenza rispetto ai relativi procedimenti autorizzatori».

nel presupposto che le misure previste non determineranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto esse saranno realizzate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dei suoi poteri di regolazione dei mercati energetici. In ordine agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.2, 2.102 e 2.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

In quel momento fu scelto - e fu fatto un errore - di ridurre le quote riservate ai cosiddetti impianti nuovi entranti, cioè quelli che sarebbero entrati in funzione negli anni successivi

provocando quindi un *vulnus* nello spirito e nella sostanza della norma europea sull'*emission trading*, che invece è basata proprio su un tentativo di rendere più efficienti i sistemi industriali in modo da ridurre l'emissione di CO2.

Il problema è vero, esiste e, se non intervenissimo, molti degli impianti nuovi entranti - penso ad esempio alla manifattura italiana - rischierebbero di fallire, perché dovrebbero pagare delle quote di CO2 che non sono in grado di pagare. Per questo con il presente emendamento proponiamo innanzitutto di non cambiare la quantità totale delle quote assegnate, per evitare che l'Europa impugni il provvedimento e determini un effetto devastante sul nostro sistema Paese: dunque la quota totale si mantiene uguale, recuperando le quote di CO2 non emesse dagli impianti nel 2009, per poterle poi concedere ai nuovi entranti. D'altra parte, nella concessione gratuita delle quote di CO2 ai nuovi entranti,

Questo è il senso del nostro emendamento. Prendo sul serio ciò che ha detto il Sottosegretario e, nel caso in cui l'Assemblea decidesse di bocciare mi aspetto che il Governo, nel più breve tempo possibile, già nel prossimo provvedimento, provi a sanare questa situazione, che nel corso degli anni che vanno da qui al 2012 continuerebbe a provocare un effetto

Signor Presidente, vorrei che lei riferisse al presidente Schifani Ieri è stato licenziato un delegato della FIOM a Pomigliano, oggi sono stati licenziati tre delegati della FIOM a Melfi. La cosa è assai grave. Chiedo che il ministro Sacconi venga urgentemente a riferire, perché se questa è la risposta ad opinioni diverse nella dinamica sindacale e nella dialettica sociale, è una risposta assai pericolosa, che porta indietro la democrazia di questo Paese di almeno trent'anni! Capisco che alcuni possano sorridere, ma quando ragazzi con famiglia vengono licenziati per motivi privi di fondamento e solo perché hanno una tessera in tasca, mi preoccuperei, anche se non fossi d'accordo con loro, anche se fossero di un altro sindacato o di un partito diverso dal mio! Credo sia una vicenda grave e che il ministro Sacconi debba venire urgentemente a renderne conto, per le sue competenze, in quest'Aula.